e finanza rappresenta forse l'atto più importante della politica economica italiana. Si tratta di definire gli andamenti dell'economia e della finanza pubblica

su entrambi i fronti: di sostegno ad una flebile crescita economica e di rafforzamento degli equilibri finanziari. Ad esso si accompagna

dell'economia e della finanza pubblica. Ora, i tre o quattro chili di carta che sono stati resi disponibili in quest'Aula sono assolutamente surreali, come ho

è attorno a 1,50, nel rapporto sul dollaro, (ricordo che al dollaro è agganciato lo yuan cinese), in termini di

all'anno per i prossimi anni. A questo si associa l'altra causa esterna, vale a dire l'ipotesi del prezzo del petrolio a 110 dollari al barile. Anche in questo caso, le evidenze di queste settimane e le prospettive di medio termine lo danno ben al di sopra di 120-130 dollari al barile. Questo significa, per un Paese come l'Italia totalmente dipendente dall'estero per il proprio rifornimento energetico, una bolletta energetica molto più alta e prospettive di impatto sui prezzi molto più consistenti. Non a caso, in questi giorni il prezzo della benzina - tra l'altro per altre ragioni

Questo modifica, se non altro in riferimento ai circa 36 miliardi di investimenti previsti, le condizioni contabili, economiche e finanziarie del Documento. La quarta, e ultima causa interna, è è che, come negli ultimi trent'anni, come è stato fatto dai Governi di centrodestra e di centrosinistra, al Ministero dell'economia non si vuole capire un concetto davvero banale, ossia l'interazione tra le manovre di finanza pubblica, che hanno a che vedere con la spesa, le entrate, il deficit e il debito, e la retroazione di dette manovre sull'andamento dell'economia reale.

C'è un andamento tendenziale, una proposta di manovra, e lì finisce la storia. La controprova - come ho detto più volte in quest'Assemblea - è che, se andate a vedere le tabelle pubblicate in questi documenti, nelle righe in fondo

è identico quando si riferisce sia all'andamento tendenziale che all'andamento programmatico, dopo l'effetto delle manovre di politica economica. È assurdo pensare che una manovra di politica economica seria, efficace nel controllo del deficit e dei saldi finanziari, non abbia alcun impatto, né positivo né negativo, sull'andamento della produzione e dell'occupazione, ossia sull'andamento dell'economia reale. Ebbene, al di là di questi quattro elementi che rendono quei dati numeri al lotto, che di

da qui al 2014 le tasse aumenteranno di 93 miliardi euro, in valore assoluto: gli italiani, da qui al 2014, pagheranno 93 miliardi di euro in più rispetto ad oggi. A che cosa serviranno questi 93 miliardi di tasse in più? Per 26 miliardi servono a ridurre il deficit pubblico a circa 45 miliardi di euro. Ciò vuol dire, poiché su questo obiettivo il Governo pone la necessità di rendere zero in quell'anno l'andamento del deficit, che

i 93 miliardi di euro di tasse in più serviranno a ridurre il deficit per 26 miliardi, lasciando comunque da definire come ridurre ulteriormente ildeficit di 45 miliardi di euro,

la spesa pubblica, per un totale di 67 miliardi. Quindi, due terzi dell'aumento delle tasse serve a coprire coprire aumenti di spesa pubblica, e un timido terzo a tagliare il deficit, lasciando l'eredità di un ulteriore consistente taglio di deficit di 45 miliardi. Ma il fatto più assurdo - signora Presidente, concludo l'intervento, è che all'interno di questo aumento di spesa pubblica di 67 miliardi vi è un aumento di spesa corrente di 48 miliardi, un aumento di interessi sul debito pubblico, sui quali non possiamo che prendere atto in riferimento all'andamento dei tassi di interesse e dello *stock* di debito, di 27 miliardi di euro e, guarda caso, una riduzione di investimenti pubblici di 8 miliardi. È evidente che la struttura di questa manovra, che ripete

che tagli la spesa corrente, riduca le tasse sulle famiglie e le imprese, aumenti gli investimenti pubblici e sostenga la crescita economica

Proprio questo contributo ampio, dialettico e costruttivo da parte sia di esponenti della maggioranza che dell'opposizione mi consente, in via di sintesi,

al combinato disposto tra gli interventi della senatrice Poli Bortone, del senatore Lauro, che ho apprezzato in modo particolare per rigore, capacità e profondità della riflessione

per cercare di innestare processi di sviluppo. Questa è la posizione che ribadiamo. Una posizione che si esprime in termini dialettici rispetto all'impostazione di un Documento, di cui sarebbe ipocrita non sottolineare un elemento. Al di là

di partecipare al cambiamento, di portare avanti il processo di modernizzazione istituzionale e sociale di cui il Paese ha bisogno. Questo è indispensabile per aprire una stagione virtuosa di mobilitazione, di impegno istituzionale, di sussidiarietà responsabile perché, com'è emerso - ripeto - dal dibattito, vi sono iniziative che, senza iscriversi al partito della spesa pubblica ma iscrivendosi al partito del cambiamento e delle riforme, si possono concretizzare per dare slancio e vitalità al sistema e mettere in campo virtuosamente quegli elementi aggiuntivi che sono indispensabili, altrimenti il ritmo della crescita è ad andamento così lento da prefigurare un percorso difficile anche rispetto alla alla prospettiva. Ciò detto, non v'è dubbio che nel Documento alcune questioni rilevanti sono da sottolineare positivamente, ad iniziare dal tema del lavoro. È importante aver ribadito l'impegno in termini finanziari a proposito degli strumenti di tutela (soprattutto degli strumenti di tutela in deroga), che in questa fase sono stati rilevanti, anche se dobbiamo avere tutti la consapevolezza che quegli strumenti sono stati importanti e lo sono ancora per l'allargamento delle tutele che implicano, ma che vanno assolutamente accompagnati, per evitare che diventino bacini di crisi, da politiche attive del lavoro che mobilitino i bacini e determinino condizioni di reinserimento nel mondo del lavoro, altrimenti rischiano di provocare sacche che in prospettiva comportano scelte di carattere assistenzialistico. È giusto aver ribadito il tracciato riformista che parte dal Libro bianco sul mercato del lavoro e che arriva fino all'esigenza di

dalle misure di carattere temporaneo a misure di carattere strutturale, innestare la riforma delle tutele, cercare di affrontare il tema dello Statuto dei lavoratori; insomma cercare di completare quella modernizzazione del mercato del lavoro che è necessaria ed indispensabile, e contemporaneamente affrontare, con grande forza e soprattutto in alcune aree del Paese, il tema dell'istruzione come leva fondamentale per intervenire sul capitale umano, a partire dalla tragedia della dispersione scolastica. Quest'ultima, soprattutto in alcune aree metropolitane del Mezzogiorno, elimina dalla possibilità di prospettiva e di futuro intere generazioni e le abbandona al rischio della criminalità, in particolare della microcriminalità organizzata. Quindi, questo tratto è sicuramente positivo all'interno del Documento, ossia il rafforzamento sul terreno del lavoro e della filiera lavoro, istruzione, ricerca, inserimento nel mondo produttivo. Ci sono altri punti significativi ed importanti che sono stati sottolineati negli interventi ai quali facevo riferimento. Mi interessa sottolineare un dato, concludendo il mio intervento. Noi abbiamo cercato di avere un approccio costruttivo rispetto al Documento, in particolare in tema di sviluppo del Mezzogiorno, non in quanto meridionali, e non per una scelta di taglio meridionalistico, ma perché abbiamo la consapevolezza che la questione meridionale e lo sviluppo del Mezzogiorno sia un aspetto d'interesse nazionale che riguarda la crescita del sistema Paese. A tal proposito, bisogna riconoscere che molto più va fatto, sia dal punto di vista della rapidità degli interventi e dell'organicità degli stessi, sia dal punto di vista della qualità e della direzione della spesa. Infatti, il Documento stesso mostra che l'impatto addizionale dell'utilizzo delle risorse comunitarie

2007-2013, ed è già il 2011. E non mi pare che il risultato dell'utilizzo dei fondi strutturali sia particolarmente significativo nelle aree del Sud. Peraltro, anche rispetto alla spesa dei Ministeri, si pone l'esigenza di un'azione di monitoraggio, di attenzione, per seguire, accompagnare e determinare le condizioni ed evitare il rischio della perdita delle risorse o del cattivo utilizzo delle stesse, quindi un luogo di cooperazione istituzionale e sociale per fare le grandi scelte nell'interesse del sistema Paese.

un risultato importante attraverso l'approvazione del nostro emendamento, che ha evidenziato due elementi, che si tengono insieme in termini di coesione nazionale. Da una parte, l'esigenza di accelerare il piano per il Sud, di renderlo concreto, di farlo camminare, di determinare le condizioni reali per l'utilizzo delle risorse, e non per la loro elencazione. Dall'altra, la consapevolezza che il progetto federalista può determinare elementi di modernizzazione e di responsabilità tali che possono contribuire, a partire da quel che nello stesso processo processo federalista è stato evidenziato, cioè la perequazione ed il riequilibrio infrastrutturale a tenere insieme questo Paese in termini unitari. Non a caso abbiamo indicato, come impegno per il Governo, di venire in Parlamento a riferire sullo stato d'avanzamento del piano per il Sud,

cui vi è stato il concorso e l'adesione dell'intero Senato. Mi sembra anche questo un fatto importante e significativo che mi porta a ribadire, ripeto, soprattutto per questo, il voto favorevole alla proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza.

per noi dell'Italia dei Valori ci sono due modi diversi per leggere e valutare l'apparente abbondanza di dati e di tabelle contenute in questo Documento di economia e finanza. Se doveva essere lo strumento programmatorio per raddrizzare l'albero storto dei conti, per indicare la strada da seguire per un risanamento del bilancio pubblico e di come questo rigore potesse essere accompagnato ad un'azione incisiva di sviluppo e di modernizzazione del nostro Paese, allora per noi è evidente che più che un pareggio di bilancio a questo Governo interessa continuare un galleggiamento di vista. Il Documento non contiene nessuna novità, nessun messaggio forte, nessuna scossa o frustata, come volete chiamarla. Tante percentuali, tanti «zero virgola» ma nessuna priorità, nessun obiettivo concreto, nessun cronoprogramma di misure efficaci, credibili, realizzabili in tempi certi. gli esempi prima degli altri che da sempre hanno rappresentato, e non solo in questa legislatura, i vostri cavalli di battaglia: la scelta del nucleare e la riforma fiscale. Sulla confusione scoppiata nel Governo dopo Fukushima, non si va al di là della falsa ipocrisia della necessità di una pausa di riflessione che, in realtà, è servita a coprire tutta la vostra paura a far sapere cosa pensano veramente gli italiani del nucleare, e non solo su quello. Quanto al fisco, il Programma nazionale di riforma si limita a proclamare un valore strategico della riforma, ma si guarda bene poi dall'impegnarsi sul dato che sarebbe stato quello politicamente più serio e più credibile, cioè i i tempi, perché il Paese reale non è più in condizioni di aspettare. Non possiamo poi non parlare dei latitanti eccellenti di questo PNR. Sul tema delle

La politica dell'energia risulta non pervenuta. Del piano straordinario per l'efficienza energetica, che doveva arrivare entro la fine del 2009, non c'è traccia. Ancora più preoccupante è l'omissione di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, anche quella promessa da tempo. Per quanto riguarda poi la ricerca e l'innovazione, la differenza abissale - che resta invariata - tra l'investimento italiano e il livello europeo si illustra da sé,

sta pesando, più che la precarietà dei conti, la precarietà di una maggioranza che si dimostra nei fatti incapace di scelte responsabili, chiare e condivise.

Non parla più alle famiglie; eppure, dopo gli spot sul *bonus*, sui quozienti, sui fattori familiari, il Governo non fa mancare occasione per enfatizzare ed annunciare a più riprese l'intenzione di rafforzare il ruolo delle famiglie. In effetti a suo modo lo ha fatto: tutti i problemi ricadono infatti sulle famiglie, dalla povertà emergente alla dipendenza dell'età anziana, dalla disoccupazione giovanile alla cura dei bambini per carenza di strutture per l'infanzia (e ne sa qualcosa anche l'OCSE). Non riuscite più a parlare ai lavoratori, dimostrando in questo modo, oltre che indifferenza, anche ingratitudine, perché sapete che non sono stati pochi i lavoratori e i pensionati che alle ultime elezioni vi hanno espresso fiducia, strumentalizzati ed ingannati dalla propaganda di chi prometteva opportunità, sicurezza e futuro per i loro figli. Ma voi pensate veramente di poter continuare a prenderli in giro, anche con l'ultima trovata di ieri dell'apprendistato a costo zero, senza risorse aggiuntive, che si aggiunge poi all'altra evanescente di un nuovo statuto del lavoro. Non riuscite più a parlare alle imprese, soprattutto a quelle del Nord. Gli imprenditori italiani hanno ragione quando dicono di essere soli, abbandonati dalla politica, lamentando le disattenzioni di un Governo e, soprattutto, soprattutto, di un Capo di Governo, con la sua ossessiva e paranoica priorità tra le priorità: la prescrizione breve per i suoi guai giudiziari. E voi che cosa offrite a questi imprenditori? Se tutto va bene, tra qualche anno, la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, che è stata presentata come il toccasana per affrontare il tema di una libertà di iniziativa economica che già c'è nel nostro Paese. Offrite poi una riforma fiscale che è tutta di là da venire, un federalismo che, se tutto andrà bene, partirà a metà del decennio, quando l'economia italiana potrebbe già essere gravemente compromessa, all'inconsistenza di una politica industriale che, dopo il fallimento dei distretti, ora comincia a parlare di reti di imprese. Ma è certo che 39 reti di imprese sono un po' pochine in un Paese che ha 4 milioni di piccole e medie imprese! Non riuscite più a parlare al Sud, al quale state offrendo solo chiacchiere, e ne sa qualcosa il Ministro dell'economia che è costretto, quando si trova al Sud, a parlare di fiscalità di sviluppo per gli investimenti produttivi come se non fosse stato lui stesso a rimuoverne pezzi consistenti tre anni fa - e, quando va al Nord, ad assicurare che saranno pagate meno tasse, con i regimi fiscali di attrattività europea, ma solo e soltanto a Milano. Non riuscite a parlare agli enti locali, ai Comuni e alle Regioni, a cui avete sottratto un punto di PIL di trasferimenti. È una prospettiva che sapete essere insostenibile, perché vedrà aumentare il numero di quei Comuni che non potranno più rispettare il Patto di stabilità e che nelle oltre 400 pagine del Documento economico si aspettavano qualcosa di più o, comunque, di avere almeno i riferimenti quantitativi dell'impatto

attraverso un maggiore collegamento tra scuola e mercato del lavoro. Il problema poi, signor Sottosegretario, è che non riuscite più a parlare a voi stessi alla vostra maggioranza, che viene tenuta in vita giorno dopo giorno incollando i contrasti e le liti tra ex azzurri ed ex aennini, correndo dietro alle richieste dei trenta denari dei Responsabili e ai malumori della Lega.

«maggiore flessibilità operativa dei nostri velivoli». In questo Governo perennemente commissariato da un socialista come Tremonti - e non sono nostre tali parole - non riuscite neppure a parlare tra voi Ministri: voi Ministri: Galan vuole arginare lo spettro di Tremonti che aleggia già su qualsiasi decisione; la Gelmini protesta sui tagli alla scuola e all'università; Maroni non accetta la sforbiciata ai conti delle forze dell'ordine; la Prestigiacomo lancia anatemi per i tagli all'ambiente. Il ministro Brunetta - che conosce bene le cose, perché lui sì che è un economista, mentre Tremonti è solo un giurista

e l'ex ministro Bondi, in un processo di disintossicazione, pubblica un libro dal titolo «La cultura è libertà». Queste sono le credenziali con le quali ci presentiamo all'Europa: ecco la credibilità di questo Governo in Europa. Ma soprattutto (ed è qui il problema di fondo): se alla vostra politica economica non ci credete neppure voi, come potete pretendere che continuino a farlo gli italiani? Queste sono le ragioni per le quali il nostro voto sarà nettamente contrario.

Signor Presidente, il 13 aprile scorso, quando fu presentato il Documento di economia e finanza, il Presidente del Consiglio ammise - con un candore che personalmente apprezzai - di non averlo letto tutto, ma promise che l'avrebbe fatto presto.

Il Documento di economia e finanza, com'è noto, ha due parti di fondamentale contenuto politico: il Programma di stabilità, che delinea la strategia per il riequilibrio dei conti pubblici nel contesto delle regole europee, e il Programma nazionale di riforma, che mette sul tavolo quali carte il Paese intende giocarsi per rilanciare la competitività e l'economia. Questo è il primo DEF che entra nel primo semestre europeo di questo nuovo impianto di contabilità. Il Programma di stabilità, a sua volta, ha due obiettivi principali. Il primo è la correzione del deficit, che nel 2010 si è ridotto al 4,6 per cento, ma che entro il 2014 dovrà arrivare al pareggio. Questo obiettivo appare difficile, perché ancora non sappiamo quanto la manovra del 2010 inciderà sul PIL e sulla crescita, che è già inferiore a quella dei nostri maggiori Paesi concorrenti. Alla fine del triennio saremo scesi all'11° posto nell'economia mondiale, in coda non solo a tutti gli

I rapporti deficit*-*PIL e debito-PIL non sono risaliti per colpa del Governo, ma a causa della crisi internazionale, che ha fatto crollare il denominatore del rapporto, cioè il PIL. Proprio per questo ora non si può pensare di raddrizzare i rapporti giocando semplicemente sui numeratori, tagliando la spesa e aumentando le tasse, quando i tagli lineari non sono sopportabili (come nel caso del FUS su cui si sono precipitosamente annullati tagli già approvati, aumentando invece le tasse sulla benzina). Bisogna agire sul denominatore, cioè sul PIL che, per

trainanti emergenti. A questo dovrebbe servire il Programma nazionale di riforma, e non a dare un'ulteriore limatina ai saldi, poiché di spesa pubblica improduttiva, in verità, ce n'è ancora un bel po' e continua a crescere, come ha ricordato il senatore Baldassarri. Il PNR deve soprattutto guardare al futuro, progettare il cambiamento strutturale dell'economia e della società incidendo sulla competitività del Paese, che nelle classifiche internazionali è scesa intorno al 55° posto, sul pieno utilizzo dei fattori produttivi, a cominciare dal lavoro delle donne e dei giovani, sulla capacità di attrarre investimenti anche dall'estero e, quindi, sull'aumento della produzione e

per la loro produttività. Quindi la crescita del Paese è l'aumento dell'impiego dei fattori produttivi e/o l'aumento della loro produttività. Di qui non si scappa. E il Mezzogiorno è esso stesso il grande fattore produttivo sottoutilizzato, al punto da consumare ricchezza nazionale, quando invece potrebbe crearne. Ed è così per tutti i grandi dualismi che segnano, come cicatrici profonde, l'economia italiana: il Nord e il Sud, il lavoro degli uomini e quello delle donne, il lavoro degli anziani e quello dei giovani. Ciascuno di questi divari è tale perché importanti risorse del Paese sono e restano sottoutilizzate. Al Sud lavora un giovane

Qualcuno spera che venga in nostro soccorso la riprese europea e mondiale? Non è così. Proprio perché il mercato è globalizzato, ad agganciare la ripresa saranno prima (e forse solo) i Paesi più competitivi che segneranno un *gap* che andrà a consolidarsi nel tempo. Non potendo competere sui costi del lavoro

un ufficio delle riforme smarrite: su uno scaffale ci sono le liberalizzazioni, ci sarà la riforma fiscale annunciata e non realizzata, la legge anticorruzione che giace da un anno in Commissione. L'unica riforma fiscale, di fatto, è il federalismo fiscale, di cui però si è un po' smarrito il senso, perché probabilmente finirà per aumentare le tasse anziché ridurle: succederà che una famiglia di reddito medio, fra addizionali IRPEF, tasse di scopo dei Comuni e aumento delle tariffe dei servizi urbani, pagherà più tasse di quante ne paghi adesso per coprire i costi di tutte le piccole IRI locali e municipali. Il liberalismo municipale deve essere anch'esso su qualche scaffale dell'ufficio delle riforme smarrite. Così come il fisco per le famiglie (il quoziente familiare o il fattore famiglia), e quello per le imprese, la fiscalità di vantaggio degli investimenti produttivi, diversa tra Nord e Sud in relazione ai diversi livelli di disoccupazione nelle aree del Paese, gli interventi a sostegno della patrimonializzazione attraverso la detassazione degli utili reinvestiti, la riduzione dell'IRAP, che invece non avviene e dà luogo quasi ad una fiscalità di svantaggio, potremmo dire, in questo momento. Queste sono le riforme che potrebbero rilanciare i consumi e gli investimenti, e spingere la crescita sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Il rigore finanziario è giusto nei saldi, lo abbiamo detto tante volte, ma andava accompagnato dalla selettività da vere riforme per la crescita. La selettività dei tagli sarebbe anche servita a finanziare le riforme quando non sono a costo zero. Invece non si è attuata una seria razionalizzazione della macchina amministrativa, non si sono ridotte né abolite le Province, non si sono tagliati gli sprechi e gli sperperi frutto di amministrazioni dissennate. Il Documento di economia e finanza era una grande occasione e meritava più attenzione: sarebbe servito al Paese e anche al Governo. Bisognava contenere il disavanzo e puntare sulla crescita non si fa nessuna delle due cose. Allora, delle due l'una: o il Governo non sa come fare a spingere su questi elementi, oppure lo sa ma evita o rimanda scelte impopolari, come si usa dire "spedisce la palla in tribuna" e rimanda la cura da cavallo a quando succederà qualcosa di diverso. impossibile tradurre in un vero progetto di riforma le molte promesse fatte, le riforme epocali, le scosse all'economia, e così via. Lo dico senza polemica, e personalmente anche con un po' di rammarico.

efficace, disse che l'economia è un *videogame* dove spuntano sempre nuovi mostri. Questo forse è uno di quelli. Sappiamo che il sonno della ragione genera mostri e, siccome ci ostiniamo a credere che il Governo sia formato da persone intelligenti e ragionevoli, il nostro consiglio è quello di svegliarsi. Però in fretta. Il nostro voto sul provvedimento

questo Documento rappresenta il primo atto del nuovo ciclo di programmazione economica e finanziaria che deriva dalla legge n. 39 del 7 aprile 2011, di modifica della legge di contabilità

Il nostro Paese oggi ha il secondo debito pubblico in Europa, il quarto debito pubblico al mondo (da pochi giorni siamo stati superati dalla Germania) per un recupero differenziale grazie alla nostra buona amministrazione, e questo per responsabilità di gestioni del passato che hanno devastato la nostra finanza. La sinistra su economia e finanza vuole sempre fare scuola agli altri eppure continua a dichiarare che il Governo non ha forza politica ed ha zero obiettivi (mi sembra di sentire una battuta famosa di un allenatore di calcio). Ricordiamo che la sinistra è quella forza che in economia ha inventato il "tesoretto" (che non c'era) con vera finanza creativa. Qualcuno ha definito il PD, alla domanda «cos'è la sinistra?» (che riporto qui amichevolmente), «come i bambini dell'asilo che sono fidanzati con le bambine dell'asilo, ma queste non lo sanno». Visto che alla sinistra piace fare scuola, forse dobbiamo aspettare che vada alle elementari e alle medie. Sempre sul tema del debito pubblico, ricordiamo anche le manovre che devono fare gli altri Paesi europei. La Francia farà una manovra di 28,3 miliardi di euro in due anni che andrà a colpire due capisaldi dello Stato francese: dipendenti pubblici e pensioni;

Queste manovre vogliono dire razionalizzazioni e contrazioni. Noi - ieri abbiamo ascoltato anche la sottosegretaria Viale - non abbiamo bisogno di queste manovre e, quindi, vuol dire che abbiamo ben amministrato in questo periodo di crisi e difficoltà. Sempre ricordando gli insegnamenti del Partito Democratico, «la sinistra italiana o si mostra credibile, affidabile e praticabile oppure resta all'opposizione». Lo dice anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il Programma nazionale di riforma è il fulcro del Documento di economia e finanza e sintetizza le azioni di riforma strutturale avviate e in fase di definizione. I punti inseriti vanno dal federalismo fiscale, alla riforma fiscale, al sostegno delle nostre imprese (soprattutto di quelle medio-piccole, che rappresentano il 95 per cento del totale delle imprese), alla sfida nell'ambito energetico con un ruolo importante delle fonti rinnovabili, all'innovazione dell'istruzione, alla riforma del mercato del lavoro, allo sviluppo delle aree deboli del Paese; infatti, siamo convinti che debba assolutamente avvenire lo sviluppo del Sud, che deve essere fatto però e prioritariamente tenendo conto della legalità e della responsabilità soprattutto degli amministratori locali. La sinistra per "punzecchiarci" ha enfatizzato la proiezione presente nel DEF sul contributo dell'immigrazione per il rientro del debito pubblico per i cosiddetti costi dell'invecchiamento. Siamo assolutamente insensibili a queste modeste provocazioni: è una semplice ipotesi ed un esercizio matematico, tra l'altro spinto fino al 2060 (ben 50 anni di proiezione). vediamo che pochi mesi di crisi in Tunisia, Egitto e Libia, rivoluzioni popolari che non siamo stato in grado di prevedere, oppure tragici eventi naturali come il sisma e lo tsunami in Giappone con gli effetti indotti, sempre che non siamo stati in grado di prevedere, hanno a cascata rilevanti effetti sulle economie mondiali, facendo saltare tutte le proiezioni. Senza poi contare e valutare i comportamenti ed i cambiamenti psico-comportamentali della società ed i possibili scenari di evoluzione. Quindi, è un semplice esercizio matematico. Sui numeri ci interessa di più vedere l'attuale spesa corrente ed in conto capitale delle Regioni. Cito alcuni esempi in relazione alla spesa corrente del 2009 in percentuale sul totale delle Regioni:

sono evidenti sperequazioni a danno del Nord; quindi, per noi la riforma più importante, di svolta, inserita nel Documento di economia e finanza, è quella federale, su cui il Governo sta camminando spedito. Noi, come Lega, saremo molto attenti, nell'elenco di queste riforme, allo sviluppo delle politiche sull'energia, alla modifica nell'ambito del lavoro e dell'istruzione, alle varie liberalizzazioni che verranno messe in atto con la logica esclusiva e prioritaria del miglior servizio al cittadino.

Il nostro «rimbalzo commerciale» è stato però molto più modesto rispetto all'area euro e alle altre economie. Vogliamo pertanto anche più semplificazione e meno burocrazia per rendere più competitive le nostre aziende: oggi per assolvere i 15 diversi pagamenti richiesti dal fisco italiano le nostre piccole e medie imprese perdono complessivamente 285 ore all'anno, sottratte alla produzione. Le riforme quindi risolveranno un fisco oggi opprimente ed una burocrazia oggi ottusa. Nel campo dello sviluppo economico e del commercio vorrei fare una breve riflessione riguardo ai cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), ai quali si aggiunge il Sudafrica, il cui emergere sulle scene economica, finanziaria e politica internazionali oramai è chiaramente un fenomeno che non è passeggero. Ci sono tre questioni nelle relazioni commerciali tra l'Italia e i BRIC.

Infine, il profilo di specializzazione internazionale dell'Italia la rende vulnerabile alla capacità dei cosiddetti BRIC di esportare beni di qualità sempre superiore anche in comparti tradizionalmente nostri. Nel DEF troviamo le proposte anche a queste sollecitazioni. Siamo tutti convinti però che il primo impegno a cui tutti noi dobbiamo puntare è la tenuta dei conti pubblici e la previsione di un abbassamento del rapporto deficit-PlL. La riduzione del debito pubblico è un impegno inderogabile. Il DEF presentato assicura questi obiettivi. Governo di continuare con decisione. I cittadini ci chiedono di cambiare questo Paese. Abbiamo bisogno, oltre alla tenuta dei conti pubblici, di rilanciare anche i consumi e di rimettere in moto l'economia e quindi di tenere al centro della nostra attenzione il lavoro.

il Conte di Cavour nel 1854 presentò un bilancio del Regno di Sardegna che prevedeva di destinare il 10,7 per cento delle spese alla realizzazione di nuove tratte ferroviarie.

e un'ulteriore diminuzione è programmata nel prossimo triennio. Può il sistema Paese reggere a una così evidente negazione di futuro? Certamente no, e per questo andrebbe cambiata l'impostazione della politica economica. L'occasione ci sarebbe, ed è rappresentata dal nuovo semestre europeo, che pone dei vincoli ma offre anche delle risorse: una maggiore disciplina di bilancio, ma con l'esplicita finalizzazione di un quadro di nuove azioni per una maggiore crescita. Vorremmo che fosse un'occasione anche per un dibattito pubblico. Oltre la malafede di alcuni propagandisti di Governo. Pochi giorni fa il ministro Sacconi ha dichiarato: «Non oso pensare cosa sarebbe stato del nostro Paese se in questi tre anni avessero governato loro», cioè noi del PD, dell'opposizione. pure, signor Ministro, pensi pure, che il pensiero è sempre utile. Vedrebbe come è stato, quando abbiamo avuto la responsabilità di Governo, cosa vuol dire avere una reputazione in Europa, saper calare, come è avvenuto in quegli anni, la spesa pubblica di 7 punti privatizzare ed aprire mercati chiusi, dettare nuove regole del lavoro senza compromettere le tutele essenziali. Avrebbe visto azione invece del presente immobilismo. Noi apprezziamo invece le parole nette con cui il ministro Tremonti nelle pagine di apertura del Documento di economia e finanza scommette sull'integrazione europea, diverse da quelle di un euroscetticismo aggressivo da lui dispensate per molti anni. Ci piacciono queste parole come non ci piacevano quelle. Sottolinea giustamente Tremonti gli effetti politici del nuovo patto che prenderà - dice il Ministro «la forma di una sistematica e sempre più intensa devoluzione di potere dagli Stati Nazione ad una nuova e sempre più politica entità europea». II problema è che negli stessi giorni altri Ministri autorevoli spargono a pieni mani un populismo antieuropeo, evocano «meglio senza questa Europa». Invece c'è bisogno di un messaggio chiaro ed univoco: scommettiamo su una buona Europa perché scommettiamo su noi stessi. L'Italia deve perciò decidere del suo futuro; i problemi li conosciamo tutti. Per l'economia reale c'è una crescita troppo scarsa, figlia di una scarsa produttività dei fattori; siamo cresciuti la metà degli altri Paesi e abbiamo perduto in due anni quasi l'intero guadagno del PIL nel decennio precedente. poco lavoro, specie per i giovani e le donne; c'è una crescita dell'inflazione e un impoverimento reale delle fasce a reddito medio. C'è infine il rischio che il nostro sistema produttivo non riesca ad inserirsi in modo adeguato nella ripresa mondiale. L'ISTAT ci segnala un eccezionale peggioramento del deficit commerciale dell'Italia. La situazione è perciò straordinaria e richiederebbe azioni straordinarie. Noi le abbiamo ancora una volta indicate, con la relazione di minoranza del senatore Morando, con decine di interventi dei colleghi del Gruppo e con una proposta di risoluzione parlamentare. Si può fare molto di più, se si vuole. Europa, stabilità, crescita, coesione sociale e territoriale sono le parole chiave della nostra proposta. Si può subito rendere il fisco più equo, premiando lavoro ed impresa, finanziandosi su evasione ed eccessivi favori del trattamento fiscale delle rendite finanziarie. Si può spendere molto meno con una totale e coraggiosa revisione del bilancio: troppe duplicazioni, troppo Stato nella periferia, troppi appesantimenti burocratici. Sono necessari semplificazione, buona concorrenza, sostegno agli investimenti in ricerca (per non lasciare sole le imprese) una straordinaria valorizzazione del patrimonio pubblico, per abbattere il debito e ricavare risorse. È necessario insomma scacciare la spesa cattiva per sostenere quella buona, quella che crea futuro, investendo sui beni comuni, sulla coesione familiare (la famiglia, così presente nelle vostre chiacchiere e così assente dalle politiche), sul capitale umano, sulla lotta alla povertà e all'eccesso di disuguaglianza, che sono enormi fattori di ritardo nella buona crescita possibile. Cosa fa invece il Governo? Non esce da una ordinaria manutenzione. Il DEF disegna un faticoso percorso di rientro dal picco di un debito del 120 per cento, figlio certo della crisi, ma anche di ritardi e sottovalutazioni da parte del Governo. Il percorso si affida però al permanere di un'elevata pressione fiscale. Si effettua il pesantissimo taglio degli investimenti sopra ricordato. Aggiungo solo un altro dato: per la missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio si dimezzano gli investimenti (questo accade nell'Italia del dissesto idrogeologico). Si programma una manovra correttiva con una riduzione ulteriore della spesa primaria di 4 punti nel triennio; obiettivo ambiziosissimo, che la maggioranza in carica non è mai stata in grado di raggiungere in passato. Viene programmata una manovra aggiuntiva di circa 40 miliardi di euro, se basterà, naturalmente; nonostante le negazioni del Governo, si prospetta oggi una manovra di 8 miliardi di euro. Il problema è - come abbiamo detto - che non si dà alcuna indicazione di come il Governo intenda raggiungere un risultato così ambizioso. Solo dopo una nostra battaglia siamo riusciti ad obbligare il Governo, come prevede la legge, ad esplicitare che metà di questa manovra (almeno 20 miliardi di euro) sarà a carico del sistema delle autonomie. Il Governo del cosiddetto federalismo pensa che il sistema delle autonomie possa essere un salvadanaio a cui ancora attingere liberamente senza nulla concordare per supplire all'incapacità di una buona gestione delle risorse dello Stato centrale. Ma è sul Programma nazionale di riforma che il Governo dimostra un atteggiamento completamente rinunciatario. Si tratta di un complesso di azioni, con una griglia di 85 azioni di riforma, molte certamente condivisibili, ma senza un'indicazione di priorità, di scadenza, di finanziamento, di effetti concreti. Possiamo dire, come ha osservato l'economista Tito Boeri, che l'acronimo PNR si traduce più propriamente nelle parole «proprio niente riforme». È del resto il Governo stesso che lo riconosce. Esso infatti stima in un modestissimo 0,2 per cento annuo il contributo alla crescita dato dal PNR. Siamo ai limiti dell'irrilevanza statistica. Ricordate la famosa scossa all'economia? L'annuncio dato dal Presidente del Consiglio il 31 gennaio: «Vogliamo portare la crescita oltre il 3-4 per cento in cinque anni,

C'è da non crederci, ma i dati presentati dicono che il Governo programma esplicitamente l'emarginazione competitiva del nostro Paese. Con gli obiettivi che si è dato resteremo negli ultimi posti nella graduatoria tra i 27 paesi per molti degli obiettivi sensibili individuati dal Consiglio europeo. Saremo ventiseiesimi su 27 per il livello di occupazione, ventiseiesimi per gli abbandoni scolastici, ventisettesimi per il tasso di laureati. Come può il Governo chiudere gli occhi? Manca nella proposta del Governo un'idea forte, la volontà di affrontare le sfide epocali. È la debolezza politica della maggioranza che lo impedisce. Carlo Cattaneo, studiando i fattori Cattaneo, studiando i fattori del primo sviluppo capitalistico dell'economia del Nord a metà dell''800 scriveva: «Non c'è lavoro, non c'è capitale che non incominci con un atto di intelligenza. Chiuso il circolo delle idee, resta chiuso il circolo della ricchezza». È proprio così: chiudete il circolo delle idee per la mancanza di un'idea politica forte su cui basare un serio confronto nel Paese e un appello alle energie migliori che ci sono e che dimostrano di saper reagire, se ben orientate e guidate. E questo è il fondamentale motivo del nostro giudizio negativo sulle proposte del Governo. *(PdL)*. Signor Presidente, non mi soffermerò sull'impianto complessivo del DEF e del

il suo rigore nella tenuta dei conti pubblici. Ma ho avuto la sensazione che tutti si siano limitati all'analisi. Tutti hanno detto perché non si cresce e perché abbiamo tenuto bene i conti pubblici. Io credo, invece, che lo sforzo del DEF, e in particolare del Programma nazionale di riforma, è quello di dire che cosa dobbiamo fare in concreto per crescere. Proverò a fare alcuni esempi. Il primo è il seguente:

appalto bandito da un ente pubblico di importo inferiore a 500.000 euro, quindi con procedura semplificata, bandito in data 9 novembre 2009, non sia ancora giunto a termine? Questo, perché c'è una serie incredibile di termini proposti dallo stesso decreto legislativo n. 163 del 2006, che impedisce, seppure all'alta dirigenza di un ente, di fare un appalto minore dopo un anno e cinque mesi dalla sua concreta proponibilità. Quando ai colleghi della sinistra dico che proporremo - come abbiamo fatto in altre occasioni - di ridurre drasticamente quei termini, di evitare che il DURC, cioè un certificato, abbia bisogno di 30 giorni e più per poter essere presentato,

delle maglie di una rete da pesca? O non è il caso che si dica anche che alcune direttive comunitarie sono eccessivamente burocratiche e costituiscono esse anche un impedimento alla crescita? Dobbiamo avere il coraggio di fare queste considerazioni, altrimenti non si può fare dell'Europa una specie di totem e dall'altra parte chiedere che si semplifichi. Ci sono situazioni che non vanno, e a testa alta vanno denunciate, proprio perché si deve tentare di riportare il nostro Paese

Il decreto per lo sviluppo economico, dicono i giornali, riproporrà la questione del cosiddetto *social housing*. Lo stesso nome, più o meno, aveva il "piano casa" da noi proposto più di un anno fa. Era il momento della crisi profonda, e tutti convenivamo che la ripresa dell'edilizia era perfettamente anticiclica e quindi necessaria in quel momento. Sta di fatto che la legge nazionale non è stata mai applicata da moltissime Regioni, perché è ovvio che ci sono leggi regionali assolutamente necessarie, ma non sono mai state emanate. Quel piano casa non è andato in porto. Quel piano casa non ha avuto i suoi effetti. Chiedo allora ai colleghi dell'opposizione per quale motivo in quel momento, mentre qui se ne riconosceva la necessità, le Regioni a conduzione dei colleghi dell'opposizione - vengo dalla Puglia, e ne sono testimone

porranno in concreto questi obiettivi e con le quali ci proponiamo di rompere le incrostazioni. Naturalmente, a questo andrà aggiunta la grande riforma fiscale, ma non mi ci soffermerò a lungo, perché in quel caso dovremo impegnarci e parlare sapendo che oggi il carico sulle imprese è praticamente insopportabile

signor Presidente, sulla tabella presentata dal Governo. Voglio dire ai colleghi dell'opposizione che bene hanno fatto a richiederla. È un adempimento di legge e quindi andava fatto. Il Governo l'ha fatto. Ma vorrei che in questa sede si riconoscesse la profonda onestà intellettuale del Governo che ha potuto dire che, per la manovra 2013-2014, non si può che prevedere una ripartizione degli oneri più o meno simile a quella precedente. Perché? Perché a mio avviso non è un esercizio intellettuale, ma una previsione fondata sulla serie storica. È del tutto chiaro che per non dire sciocchezze, che avrebbero potuto far comodo al Governo, abbiamo fatto una una previsione seria. È altrettanto chiaro però che siamo coscienti che il cambiare delle condizioni, ad esempio una crescita più sostenuta, potrà dare a quelle manovre non solo una diversa entità ma anche una diversa proporzione.

a settembre saranno determinate in sede europea le manovre per il 2013-2014; la previsione nazionale dice che avremmo dovuto determinarla già oggi, in anticipo sulle scadenze europee e il nostro Governo lo ha fatto. Mi pare un modo serio di rispettare un'esigenza giusta,

siamo d'accordo con le posizioni della Presidenza a prescindere, Commissione affari esteri del Senato ha deliberato all'unanimità una moratoria della revisione del piano di razionalizzazione decidendo di approfondire e di fare un'apposita indagine conoscitiva. Mi pare contrastare con l'*iter* dell'indagine conoscitiva voler discutere prima ancora che questa sia finita. A me sembrerebbe opportuno optare per

La moratoria richiesta era tesa proprio ad aspettare il risultato e l'esito di questa indagine, che dovrebbe fare delle proposte, secondo me, più costruttive e interessanti. Era su questo che c'è il consenso: cioè, c'è confusione in quanto detto dal collega Divina.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 13 aprile i presentatori hanno illustrato le mozioni. Comunico che è stato presentato un ordine del giorno unitario, sottoscritto dalla senatrice Finocchiaro e dagli altri firmatari delle mozioni,

un ordine del giorno condiviso su un tema particolarmente importante, che ha visto i Gruppi parlamentari, ma in particolare l'opinione pubblica ed i titolari di queste concessioni balneari, impegnati

Colleghi, la prossima volta sospendo la seduta. Vi ho già detto che, tra iscritti a parlare e dichiarazioni di voto ci sono due ore di lavoro circa. L'importanza di questo ordine del giorno è dovuta al fatto che, come si dice nelle stesse premesse, abbiamo 28.000 concessioni rilasciate per finalità turistico-balneari con strutture amovibili e circa 1.000 pertinenze demaniali o manufatti inamovibili di proprietà dello Stato. Peraltro, occorre ricordare che l'Italia, con i suoi 7.458 chilometri di costa, ha una specificità particolare nel contesto europeo,

lo stesso Ministero del tesoro si è reso interprete di tale esigenza e della specificità di queste concessioni balneari. Ricordiamo peraltro che le imprese che operano sul demanio marittimo dispongono delle concessioni, perché si verifica un effetto indotto che coinvolge alberghi, campeggi, ristoranti, imprese nautiche eccetera. Quindi, una serie di imprese che danno lavoro e occupazione a migliaia e migliaia di persone.

questo ordine del giorno o no? Perché non è un obbligo, come se si dovesse fare un tema. Questa è stata la scelta definita nel calendario, questa è la discussione che c'è. Vorrei che il senatore Cursi potesse illustrare per tutti questo ordine del giorno. l'Italia presenta una sua particolarità nelle concessioni balneari, e tale tipicità l'ha resa anche famosa in tutto il mondo, perché alcune spiagge vengono citate negli annuari del turismo internazionale. D'altra parte, non mi sembra che la Francia, la Spagna e la Grecia, dove si registra la diffusione di queste pratiche, presentino caratteristiche di questo tipo. Occorre quindi immaginare di difendere fino in fondo queste piccole e medie imprese, che tra l'altro rientrano nella accezione dello dalla Commissione europea, riferito proprio alla dimensione di tali aziende. Ricordiamo a tutti che proprio attraverso il lavoro fatto in questa Aula e nelle Commissioni siamo riusciti quanto meno a prorogare le concessioni balneari fino al 31 dicembre 2015.

Vorrei ricordare, peraltro, che il decreto di attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, approvato nel maggio dello scorso anno, ha devoluto alle Regioni competenze in materia di gestione delle concessioni demaniali marittime e qualche Regione si è mossa in questo senso: anche questo è un fatto estremamente importante. L'approvazione del cosiddetto federalismo demaniale ha peraltro sollecitato l'urgenza di costruire un nuovo quadro normativo per l'intero settore, richiesto in data 7 ottobre 2010 dalla Conferenza delle Regioni. Anche questo è un impegno dal quale non possiamo tirarci fuori e per il quale anzi abbiamo sollecitato il Governo, nella persona sia del ministro di Fitto, sia del ministro del tesoro Tremonti. Che l'argomento fosse particolarmente sentito, non solo dai titolari ma anche dal Parlamento e dalle Commissioni, emerge dal fatto che nei mesi scorsi,

(non solo balneari, ma anche di altre attività) e dal confronto con esponenti regionali, comunali e provinciali suggerimenti e proposte che potessero andare incontro alle esigenze delle aziende.

per sensibilizzare l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste dalla "direttiva servizi", proponendo alla Commissione europea modifiche volte a escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dalla "direttiva servizi"». Il tema fondamentale, convincere l'Unione europea che la specificità delle imprese italiane è tale e tanta da dover necessariamente garantire l'esclusione dalla direttiva Bolkestein, così come è avvenuto fino ad oggi. Ci auguriamo che, con il sostegno del ministro Fitto e del Ministro del turismo,

Governo «a valutare ogni più opportuna iniziativa al fine di non penalizzare il settore turistico-balneare e relativi livelli occupazionali». Da ciò discende l'esigenza di garantire

della parte I del Codice della navigazione, con particolare riguardo all'articolo 49, nella parte in cui esclude ogni indennizzo per il concessionario in caso di devoluzione delle opere allo Stato». Al riguardo vorrei ricordare che il protocollo di intesa

«a proseguire nell'impegno di raggiungere un accordo tra Esecutivo, Regioni e rappresentanti delle organizzazioni del settore turistico-balneare sulle problematiche legate alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, di un quadro legislativo per il settore fondato su una durata delle concessioni proporzionata all'entità degli investimenti e che salvaguardi gli investimenti effettuati dalle imprese stesse .

il percorso da fare, per arrivare fino in fondo e avere la possibilità di giungere quanto prima alla definizione di un quadro legislativo che salvaguardi il nostro Paese, le concessioni balneari e quindi le piccole e medie imprese che sono un patrimonio importante del

mettere a punto una legislazione quadro, è anche quello di mettere delle regole, perché in questo settore ormai la *deregulation* è fin troppo diffusa in molte parti del Paese.

e invito il Sottosegretario Mantica a trasmetterlo a chi di competenza. Dal momento che si svolgono così poche discussioni che riguardano temi concreti, e il turismo in particolare, sarebbe stato molto interessante che il Ministro - visto che abbiamo un Ministro - fosse presente alla discussione. Ad ogni modo, abbiamo un autorevole Sottosegretario, che trasmetterà al Ministro quanto qui discusso.

girato l'Italia - per così dire - e abbiamo conosciuto là dove operano, nei loro territori, gli operatori del settore balneare. Sottolineo che si tratta di aziende a forte tradizione e a forte caratterizzazione locale e nella maggior parte dei casi di strutture gestite a livello familiare, che riguardano centinaia di migliaia di persone.

proposta turistica tra le più importanti d'Italia, vi sono 480 chilometri di costa. Abbiamo svolto un grande lavoro,

previste dalla direttiva servizi (Bolkestein), che effettivamente rischia di mettere in ginocchio questo importante pezzo dell'economia italiana, ad escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo, in virtù della specificità del settore, della rilevanza degli investimenti materiali ed occupazionali e dell'unicità del settore a livello europeo. In tal modo, si riuscirebbe a non penalizzare il settore turistico-balneare

pagano l'IVA più alta nel settore, al 20 per cento. Quindi, anche con la presentazione di alcuni testi di legge, vorremmo provare a continuare a svolgere questo lavoro.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, anche oggi ci apprestiamo a trattare una questione che riguarda l'istituzione Europa e che incide, ancora una volta, in modo negativo sul nostro Paese. L'Unione europea, purtroppo, ci sta dimostrando spesso incapacità nell'affrontare temi importanti che riguardano da vicino tutti noi. Pensiamo, ad esempio, a come l'Unione europea si è comportata in merito alla gestione dei flussi migratori verso le nostre coste dopo l'implosione dell'intera area del Maghreb. In tale occasione in tanti ci siamo chiesti: dov'è l'Europa con le sue istituzioni? Qual è la sua politica? E ci meravigliamo dell'assenza dell'Europa nel sostenere i suoi Stati membri nel momento di necessità, come quello dell'emergenza umanitaria che è stata affrontata in totale solitudine dal nostro Governo. E qui, cari colleghi, non posso che condividere anche le parole del cardinal Tarcisio Bertone che, in quel frangente, ha espresso in merito all'emergenza la delusione della Chiesa nei confronti dell'Europa. Mi sono soffermato inizialmente sul contesto generale poiché è l'ulteriore riprova di come questi accadimenti abbiano fatto diminuire e di molto la fiducia degli italiani nell'istituzione europea, quell'istituzione che non è nemmeno riuscita a decidere di fondare la sua esistenza su quelle radici cristiane che, anche storicamente, non possono essere sconfessate. Penso anche che sia doveroso da parte nostra far capire a chi ha ruoli di rappresentanza di quell'istituzione e proviene da altre Nazioni, come ad esempio la Francia, la Germania e l'Inghilterra, che non esiste un'Europa di serie A ed una di serie B, anche perché se così fosse, per storia, cultura, ingegno e valori positivi noi saremmo di gran lunga i primi in classifica, ma che deve affermarsi, invece, come anche ricordato dal presidente Napolitano, un'Unione europea solidale, scevra da egoismi. Da un'Europa che si divide sui valori fondanti ad un'Europa che dà il senso di una mancanza di azione politica comune, ad un'Europa che, invece, fa valere con forza le sue prerogative burocratiche e di controllo sui mercati degli Stati membri e che incide in modo particolare su quelle attività che caratterizzano il nostro Paese per la qualità dei servizi e dei prodotti. Non possiamo dimenticare le battaglie che abbiamo sostenuto per far capire all'Unione europea l'importanza del *made in Italy*. Tutti noi siamo orgogliosi di questo *made in Italy* e abbiamo legiferato per aiutare le imprese a far rimanere le produzioni nel nostro Paese e poi, invece, spesso dobbiamo scontrarci con i provvedimenti delle istituzioni europee che un giorno ci mettono in difficoltà sui prodotti agroalimentari, un altro giorno non riconoscono l'importanza e dunque non tutelano le nostre aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature, sino ad arrivare alla ormai famosa direttiva Bolkestein che vuol cancellare in un colpo solo una tipicità che è propria del nostro turismo, quella degli stabilimenti balneari che danno un servizio di spiaggia ai tanti turisti che soggiornano lungo le nostre coste. Nel 2008 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione mettendoci in mora. Ciò ha causato l'abrogazione di quel diritto di insistenza previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione, che rappresentava il principio su cui fondare la continuità dell'impresa balneare. Nei mesi scorsi, insieme al collega Baldini, promotore di quella legge che aveva stabilito il rinnovo automatico delle concessioni demaniali per i balneari, abbiamo seguito da vicino gli sviluppi della situazione e ci siamo adoperati per venire incontro alle esigenze espresse dalle associazioni di categoria, anche con la presentazione di alcuni emendamenti al decreto milleproroghe. Il Governo, a sua volta, con senso di responsabilità ed in modo efficace, ha inserito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, quel comma 18 dell'articolo 1 che ha permesso alle concessioni con finalità turistica ricreative di ottenere una proroga della loro durata sino al 31dicembre 2015. Ma la cancellazione del diritto di insistenza e la prossima cancellazione anche dell'automaticità del rinnovo non fa dormire sonni tranquilli agli esercenti gli stabilimenti balneari che vedono a rischio la propria esistenza ed il lavoro di circa un milione di addetti tra impiego diretto ed indotto. Oggi più che mai queste persone vivono nell'incertezza più assoluta. Vorrei cogliere l'occasione anche per sottolineare l'esclusione dalla proroga al 2015 di quelle concessioni demaniali marittime per usi e finalità diverse da quelle turistico-ricreative. In particolare, le imprese che insistono sulle aree portuali non godono più di alcuna tutela. Mi riferisco, nel caso specifico, ad attività che spesso sono artigianali, come piccoli cantieri navali o magazzini legati alla pesca e alla commercializzazione dei prodotti ittici. La direttiva europea ha causato e sta causando anche la paralisi del settore, che, non vedendo un futuro chiaro, non investe nell'impresa e deve riscontrare una mancanza di sostegno finanziario degli istituti di credito, che in questo contesto non possono contare sulla stabilità delle aziende stesse.

È comunque indispensabile giungere ad una norma transitoria di lungo periodo, che garantisca i concessionari attuali ed i loro investimenti. Cari colleghi, questo settore rappresenta circa 30.000 aziende in Italia, aziende che sono quasi sempre a conduzione familiare; aziende e dunque famiglie che hanno sostenuto negli anni investimenti cospicui per dare un servizio sempre migliore e di qualità al cliente. Ebbene, la direttiva europea in questione vorrebbe far sì che il lavoro di decenni di queste imprese venga messo in vendita all'asta senza riconoscere loro né il valore commerciale né il valore degli investimenti, così che un'impresa concessionaria dall'oggi al domani si ritroverebbe spogliata del lavoro di una vita. Non vorrei che questa decisione sia frutto di logiche che intendono favorire grandi gruppi o comunque altri soggetti provenienti chissà da dove e che poco o nulla conoscono della nostra realtà. Non dobbiamo permettere che venga meno la forza di un settore che sino ad oggi si è contraddistinto per quella peculiarità tutta italiana che fa del servizio in spiaggia, inteso anche come ristorazione ed intrattenimento, una eccellenza del turismo del nostro Paese. Non vorrei in definitiva che sia venuto in mente a qualcuno di sacrificare questo settore per favorire interessi economici esterni al nostro Paese. Non dobbiamo, cari colleghi, permettere che ciò avvenga, ma sono comunque fiducioso del lavoro che il Governo sta portando avanti per difendere gli interessi degli operatori e credo che questo nostro ordine del giorno, che ci apprestiamo a votare, segni un passo determinate per supportare le iniziative e gli impegni che il Governo stesso andrà ad assumere. Per chi, come me, proviene da una realtà turistica importante delle Marche (Porto Recanati, città dove sono stato vice sindaco e assessore al turismo e alla cultura per dieci anni) è facile capire come in questo momento sia indispensabile sostenere le richieste degli stabilimenti balneari. Altrimenti, ci costringeranno a perdere un pezzo importante dell'economia prodotta dal settore turistico. Penso, infine, che sia un dovere anche degli italiani che oggi siedono nel Parlamento europeo attivarsi in modo deciso nei confronti di una direttiva che penalizza fortemente il nostro settore turistico, per far capire che non possiamo e non vogliamo inchinarci a decisioni che hanno l'unico obiettivo non dichiarato di destabilizzare il settore turistico del nostro Paese. La Bolkestein è una direttiva che finge una liberalizzazione del mercato, ma che in realtà avrebbe l'unico effetto di mettere a rischio il lavoro di 30.000 famiglie italiane. Per questi motivi, ci opponiamo ad essa con forza e saremo al fianco del Governo, che siamo certi si adopererà a tutela degli interessi dell'intero settore turistico-balneare. Agli amici delle aziende coinvolte dico: non siete e non vi lasceremo soli in questa battaglia, una battaglia che non è solo la vostra, poiché rappresenta una sfida lanciata all'intero sistema turistico italiano.

In un momento in cui si parla tanto di amore per l'Europa, di difesa dell'Europa, di euroscetticismo, più o meno, io credo che sia davvero difficile comprendere come qualcuno in Europa non abbia potuto tener conto di una specificità dell'Italia,

con questa direttiva, essi vengono messi sul lastrico. Il primo risultato è che non accedono più a nessun credito e che non hanno più nessuna intenzione di intervenire con investimenti all'interno delle proprie aziende. Il che significa degrado, scarsa qualità del turismo e dei servizi. Mi domando come sia possibile non immaginare che l'Italia ha una realtà turistico-balneare completamente diversa da quelle esistenti nelle

onorevoli colleghi, rappresentante del Governo nella consapevolezza che spesso mozioni e ordini del giorno appartengono un po', calcisticamente parlando, ad un girone consolatorio,

per un documento che non poteva non essere unitario se voleva in qualche modo raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva. Come hanno sottolineato anche i colleghi che mi hanno preceduto, in quest'ordine del giorno si parla molto di Europa, più di quanto le parole scritte possano far pensare.

un contenzioso tra l'Italia e il resto dell'Europa, quanto quello di provare a fare la fatica della politica. C'è un deficit di politica vero e grande dentro l'Europa, che forse fa assumere provvedimenti, atteggiamenti e iniziative che non sono sufficientemente atti politici, talvolta peccando di burocrazia, qualche altra di presunzione.

Penso che l'Europa stia ripensando un po' al significato e al valore della piccola impresa. Pensare in piccolo potrebbe sembrare oggi qualcosa di più significativo di quanto era apparso ieri, in un tempo in cui la crisi, forse, non aveva fatto ripensare ad alcuni passaggi. Allora, nella consapevolezza che questo atto ha il suo valore nell'essere unitario e il suo limite - credo - nell'arrivare dopo, sempre calcisticamente parlando aggiungerei: *por *Por què* non riusciamo ad arrivare per tempo? Forse perché quel deficit di politica non ci aiuta in questo? Forse perché l'autorevolezza anche del nostro Paese non cresce nella misura giusta? Può essere anche questo, però mi sembra che oggi si compia comunque un atto molto buono e utile alla politica di questo Paese, e anche a quella dell'Europa. È per questo, credo, che va sostenuto con grande forza. Ci sono motivi di verità nella direttiva europea. Ci sono motivi di saggezza in quanto è

Signor Presidente, il documento in esame dà voce alle tante piccole realtà locali del settore turistico-ricreativo che oggi rischiano di essere tagliate fuori dal mercato, con ricadute importanti sullo sviluppo del settore e sull'occupazione. Il turismo, infatti, è un settore strategico per l'economia del Paese ed in particolare, visto che siamo a ridosso dell'inizio della stagione estiva, l'industria balneare rappresenta un'eccellenza a livello internazionale del turismo nazionale. Basti pensare che la stessa esprime circa un terzo della ricchezza prodotta dall'intero comparto turistico. Queste piccole imprese balneari, per lo più gestite a livello familiare, sono depositarie di tradizioni che hanno radici lontane, le quali sono state determinanti per il loro sviluppo, facendo di conseguenza raggiungere al comparto un buon grado di competitività. Sul territorio sono presenti circa 30.000 aziende che occupano nel periodo estivo non meno di 300.000 persone, senza contare le persone impiegate nell'indotto. Non possiamo quindi pensare di poter procedere ad una revisione della normativa vigente - come richiesto dall'Europa - trascurando le ricadute che questa avrebbe sul settore. Fino ad oggi, infatti, le strutture turistico-ricreative hanno potuto contare su una normativa relativa alle concessioni certa e univoca, che prevede il rinnovo automatico delle stesse di sei anni in sei anni e così via. Tale quadro normativo ha permesso alle aziende balneari di pianificare nel tempo importanti investimenti nelle strutture, con ricadute positive sui territori interessati. I risultati fino ad oggi raggiunti rischiano di essere vanificati dalle posizioni assunte in materia dall'Unione europea. La stessa infatti ha aperto, nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla direttiva servizi, la quale comporta la messa all'asta delle concessioni stesse. Il ricorso alle aste avrebbe un impatto negativo sulle attività svolte dalle piccole imprese, incidendo sulla vita di circa 60.000 famiglie e su un indotto che conta oltre 400.000 persone che dall'oggi al domani potrebbero trovarsi senza lavoro. Il clima di incertezza che si sta creando nel settore avrebbe come prima conseguenza quella di scoraggiare gli imprenditori a continuare ad investire nelle strutture turistico-ricreative e questo si tradurrebbe quasi certamente in una drastica riduzione della qualità dei servizi balneari offerti ai consumatori, oltre che in un impoverimento del turismo nei territori locali. Per le ragioni appena illustrate viene sollecitato il Governo ad intervenire affinché vengano salvaguardate le peculiarità delle imprese che operano nel settore turistico-ricreativo. In tal senso, è necessario sensibilizzare l'Unione europea ad individuare per le imprese balneari italiane soluzioni diverse rispetto a quelle previste per le analoghe imprese europee con riguardo all'applicazione della direttiva servizi e nello stesso tempo arrivare il prima possibile alla definizione di un quadro normativo certo e univoco per il settore, sul quale crediamo che le Regioni possano dare un contributo importante per il fatto che le stesse, oltre ad avere specifiche competenze in materia, da ultimo rafforzate con il decreto attuativo del federalismo demaniale, sono molto vicine alle realtà locali e per questo riescono ad interpretare in modo migliore le problematiche del settore.

fatto. Credo che oggi, con la presentazione di questo ordine del giorno unitario, abbiamo dato un bell'esempio di serietà e responsabilità politica nei confronti di tutte quelle imprese che operano sul demanio marittimo e che si trovano attualmente a dover affrontare, oltre all'incertezza economica derivante dalla crisi in corso, anche e soprattutto l'incertezza normativa che riguarda la loro operatività destinata ad incidere pesantemente sulla loro stessa sopravvivenza. Nel contempo, abbiamo lanciato al Governo un messaggio forte e chiaro affinché siano presi quei provvedimenti necessari e indifferibili per tutelare un settore fondamentale per tutto il comparto turistico e per l'economia dell'intera Nazione e che sono sostanzialmente tre: uscita dalla procedura di infrazione, esclusione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo dalla direttiva servizi, riordino di tutta la materia delle concessioni demaniali marittime con un'apposita legge quadro nazionale. Ci auguriamo dunque che il Governo recepisca le istanze del Parlamento a partire dal decreto sviluppo e si attivi concretamente per tutelare un sistema di eccellenza come quello della balneazione attrezzata in Italia e consenta alle 30.000 aziende di svolgere il proprio lavoro e di effettuare con la dovuta serenità gli investimenti necessari per conservare e migliorare una peculiarità derivante da oltre 100 anni di storia, unica in tutto il panorama europeo.

conciliabili con l'interesse pubblico, sempre sotteso ad una proprietà demaniale. Infatti, se vi una proprietà demaniale vi è un interesse pubblico che deve essere tutelato, anche laddove quel bene quel bene demaniale sia fruibile da privati, che possono sfruttarlo come una risorsa di grande rilievo economico sia per se stessi, come imprenditori, sia per la collettività che, come in questo caso, ne fruisce. Quindi io mi auguro che questa particolarità assoluta, che non è stata evidentemente fatta presente nelle sedi opportune, venga oggi messa in primo piano, sia a livello di Parlamento che di Commissione e Governi europei, perché si tratta di una situazione

l'esperienza quotidiana ci dimostra. Credo che al riguardo occorra fare una giusta riflessione e tutelare in seconda battuta - ma mi auguro che sia possibile una deroga totale

a mio avviso fino ad oggi hanno offerto un servizio di livello eccellente e dei prezzi sostanzialmente contenuti. Penso che sfasciare questo meccanismo rappresenti un danno per l'intera collettività nazionale e anche per la realtà europea.

spiegare l'assenza del ministro Brambilla e questo mio ingrato compito di interessarmi di situazioni balneari. Il ministro Brambilla è al Consiglio dei ministri dove si discute il programma di sviluppo, nell'ambito del quale c'è un rilevante settore Per quanto riguarda il contenuto della discussione, quindi il documento che andiamo ad approvare,

La materia - com'è stato dimostrato nella discussione - era particolarmente delicata riguardando un settore di imprese che operano sul demanio marittimo, che sono molto preoccupate dal cambiamento del sistema, che - voglio ricordare - è regolato da una legge fondamentale di sessant'anni fa, in quanto è fondato ancora sul codice della navigazione del 1942, imperniato di per sé su di un regime di sostanziale rinnovo automatico del titolo concessorio, fino ad arrivare a un regime concorrenziale in linea - e qui viene il problema - con i princìpi di liberalizzazione e di trasparenza sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione europea. L'attuale situazione delle imprese del turismo balneare, la cui legittima aspettativa è di poter contare su di un orizzonte temporale sufficientemente lungo per poter ammortizzare gli investimenti, in taluni casi anche di importo elevato, è stata incisa dall'abrogazione del diritto di insistenza, cioè dalla preferenza accordata, nel caso di più domande di concessione, al soggetto che sia già titolare delle concessioni in scadenza. Il contenuto è stato condiviso sia in sede nazionale (il parere favorevole delle Regioni è stato acquisito nel corso della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni), sia in sede europea, con la Commissione europea, in particolare per quanto riguarda la proroga delle concessioni in essere in modo da preparare il settore all'apertura alle regole di concorrenza. Tuttavia (qui c'è la preoccupazione), in sede di conversione del decreto-legge milleproroghe del 2009, un emendamento allora approvato nel passaggio alla Camera dei deputati, attraverso il richiamo a norme precedenti, ha reso non più certo il termine ultimo di proroga delle concessioni che, nel frattempo, il Governo aveva concordato con la Commissione europea al 31 dicembre 2015. Ne risulta che la formulazione della legge di conversione non ha consentito di superare la procedura di infrazione europea. Vale la pena di ricordare al riguardo che la Commissione europea, constatato che il testo della legge di conversione non si conformava a quanto richiesto nella lettera di messa in mora del 2009, ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora complementare, la n. 2010/2734 del 15 maggio 2010. Nella lettera si chiariva che il mantenimento della preferenza per il concessionario uscente poteva far venir meno anche la disponibilità della Commissione europea a non contestare la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2015, dato che abrogazione del diritto di insistenza e regime transitorio costituivano per la Commissione europea un unico pacchetto negoziale. Per una esauriente esposizione della problematica relativa alle concessioni demaniali marittime, è opportuno rammentare che anche la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie leggi regionali che avevano prorogato il termine di durata delle concessioni. Per altro verso, il contrasto della normativa italiana con il diritto dell'Unione europea ha comportato la non applicazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, Infine, è intervenuto il Governo con il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, volto a conferire il demanio marittimo ed il patrimonio disponibile dello Stato al patrimonio delle Regioni e degli enti locali. Per conformarsi definitivamente agli obblighi dell'Unione europea, il testo del disegno di legge comunitaria 2010, approvato dal Senato lo scorso 2 febbraio 2011 ed attualmente in esame alla Camera dei deputati, è suscettibile di far venir meno l'incompatibilità con il diritto dell'Unione. La chiusura della procedura di infrazione è considerata dal Ministro del turismo la condizione imprescindibile per passare alla seconda fase, cioè alla disciplina *ex* *novo* della materia delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.

Le amministrazioni interessate hanno già tenuto numerosi incontri al fine di addivenire all'intesa, di cui alla detta disposizione, nell'ottica di una reciprocità di impegni da parte del Governo e delle Regioni nell'ambito delle rispettive legislazioni. Nel contempo si è cominciato a prefigurare le questioni da disciplinare mediante uno schema di legge quadro per l'intero settore. Tali questioni in particolare concernono: una congrua durata delle concessioni (da un minimo di 12 anni a un massimo di 30 anni) in ragione della piena valorizzazione delle aree demaniali e dell'entità degli investimenti; la modalità di affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei Trattati europei e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ma ovviamente rispondenti anche ai princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento. In tutto il percorso sopra ricordato il Ministero del turismo ha intrattenuto frequenti contatti con le organizzazioni di categoria delle imprese che operano sul demanio marittimo (alberghi, campeggi, ristoranti, stabilimenti balneari, C'è piena consapevolezza da parte del Ministro del turismo sulla necessità di dare risposte atte a rassicurare le imprese turistiche, che si trovano da tempo ad affrontare, oltre all'incertezza economica, dovuta al ciclo sfavorevole, anche una una evidente incertezza normativa, derivante dalla procedura d'infrazione europea e dalle pronunce del giudice amministrativo. In questo contesto non si mancherà di esplorare in sede europea la praticabilità di una normativa transitoria tra vecchio e nuovo regime delle concessioni demaniali marittime a finalità turistica, che tenga conto dell'applicazione per oltre mezzo secolo del cosiddetto diritto di insistenza senza che da parte della Commissione europea siano state sollevate obiezioni.

del turismo, si impegna ad esplorare in sede europea ogni azione atta a rappresentare la specificità del settore balneare, sicuramente caratterizzante il nostro comparto turistico, ribadendo tuttavia l'imperiosa necessità di non frapporre altro tempo alla chiusura della procedura d'infrazione, e che il Ministro del turismo è altresì impegnato, tenuto conto del passaggio ad un nuovo regime concorrenziale, un nuovo regime concorrenziale, a verificare la possibilità di concordare in sede europea un regime transitorio fondato sulla tutela del legittimo affidamento degli attuali operatori del settore. Il Ministro del turismo ribadisce l'impegno a rappresentare in sede di Unione europea la specificità del settore turistico-balneare italiano e altresì a verificare, di concerto con gli altri Ministri interessati, la modifica della disposizione del codice della navigazione richiamata. Tale attività sarà proseguita in leale collaborazione con le Regioni, come abbiamo fatto finora, e con la partecipazione di tutti i rappresentanti delle categorie interessate. È ovvio quindi, signor Presidente, che il Governo, nel ringraziare i parlamentari per il lavoro svolto e per il risultato conseguito, accoglie l'ordine del giorno.

onorevoli colleghi, nella scorsa seduta dedicata a questo tema, in sede di illustrazione delle mozioni, è emersa con chiarezza una condivisione trasversale sulla necessità di sostenere il settore turistico balneare, pur con alcune diversità nei dispositivi. Il 5 aprile scorso i balneari italiani, provenienti da tutta Italia, si sono dati appuntamento a Roma, in piazza Navona, davanti al Senato, non tanto per protestare, quanto per testimoniare con forza il timore, il dissenso e la frustrazione nel vedere che, nella quasi totale indifferenza delle istituzioni, si lascia che, a partire dal 2016, possano andare all'asta le concessioni delle spiagge, e con queste, indirettamente, le imprese costruite in anni di lavoro. Queste imprese chiedono di avere la certezza che il Governo italiano, non solo non le abbandonerà, ma saprà invece individuare percorsi e strumenti di salvaguardia da portare con forza all'attenzione delle competenti sedi europee. Ci è sembrato dunque un atto dovuto affrontare questo problema, innanzitutto per dare un segnale in controtendenza rispetto a quanto è stato fatto finora. C'è chi, giustamente, ritiene che il Governo non abbia difeso efficacemente in Europa il sistema balneare italiano (forse dandolo per scontato), rischiando così davvero di perdere il valore e la specificità che lo contraddistingue. È difficile, d'altronde, non pensare che per il Governo il turismo balneare sia poca cosa. Basta guardare le immagini del nuovo video lanciato dal Governo per il turismo nella «Magica Italia», in cui si resta allibiti dinanzi alla totale scomparsa del valore del mare e delle spiagge italiane, dimenticando totalmente località come la costiera Sorrentina, la costiera Amalfitana, Viareggio, Taormina, Portofino, Rimini, il Gargano e moltissime altre ancora, che hanno reso famosa e conosciuta l'Italia nel mondo. Ad avvalorare la sensazione di disinteresse nei confronti del settore, vi è poi anche la questione dell'intesa redatta dal Ministero per gli affari regionali, in data 21 dicembre 2010, che disattende totalmente la richiesta avanzata dalle organizzazioni. Quello che chiedevano gli addetti ai lavori era di produrre una necessaria disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale, che non potrà che avere forza di legge quadro, così come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 12 maggio 2010, che, in materia di concessioni demaniali marittime, ha affermato l'esclusiva competenza statale. La stessa cosa aveva chiesto la Conferenza delle Regioni in data 7 ottobre 2010. È evidente, invece, che lo strumento dell'intesa istituzionale non è quello più adatto ad affrontare questa emergenza. Allo stato attuale, pare dunque più che evidente che il Governo faccia fatica a trovare soluzioni per risolvere la problematica indicata. Abbiamo concordato, quindi, sulla proposta di lavorare ad un testo unitario perché sarebbe stata un'occasione mancata non arrivare, su un tema del genere, ad una grande convergenza. Ed ho apprezzato anche la risposta che ci ha dato il Sottosegretario. Quello che è emerso, dunque, su questo fronte, è un duplice ordine di esigenze cui ci siamo sentiti chiamati a dare adeguata e legittima risposta: da un lato, l'obbligo per lo Stato italiano di non perdurare nell'inadempimento ad obblighi comunitari e nella insensata reiterazione di periodi di *prorogatio* del regime antecedente l'ingresso della direttiva servizi; dall'altro, la necessità, per gli operatori di mercato, di usufruire di un quadro normativo stabile e serio che, conformemente ai principi della direttiva comunitaria, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare senza traumatiche soluzioni di continuità nell'attività degli operatori, sia nel breve che nel lungo periodo, oltre che nel periodo transitorio. È di tutta evidenza quale gravissimo danno si creerebbe per l'economia del nostro Paese mandando via 30.000 piccoli imprenditori - e le famiglie che ci sono dietro - dalle loro aziende costruite con tanti sacrifici, anche di diverse generazioni, generando così, oltre oltre all'evidente danno economico per chi ha investito tutto confidando sulla certezza che veniva assicurata dall'impianto normativo italiano, una situazione di grave precarietà in un settore cruciale per l'economia italiana. Non possiamo dimenticare, infatti, che le imprese turistico-ricettive hanno mantenuto livelli occupazionali accettabili anche durante la crisi economica che ancora non ci siamo lasciati alle spalle. Senza dubbio, però, è per noi prioritario che si chiuda la procedura di infrazione con l'Unione europea e che, qualsiasi iniziativa si intenda avviare, essa sia compatibile con l'ordinamento comunitario. Come vi abbiamo in più occasioni ricordato, non si può scegliere, di volta in volta, se essere o meno membri dell'Unione europea; non si può entrare ed uscire sulla base delle proprie convenienze di politica interna. Siamo nell'Unione europea ed è in questa sede che si deve affrontare la questione. Questo è principalmente quello che abbiamo voluto ribadire con le nostre proposte in questo testo: la necessità di agire, in sede comunitaria, per sensibilizzare l'Unione europea sulle peculiarità che caratterizzano le imprese del settore turistico-balneare in Italia e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste dalla cosiddetta direttiva servizi. Sta a voi ora proporre alla Commissione europea modifiche volte o ad escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dalla direttiva servizi rimanendo all'interno dei limiti della stessa direttiva, prevederne una diversa applicazione. Solo in tale quadro - lo ripeto - è possibile trovare la soluzione non solo migliore, ma legittima e soddisfacente nell'interesse dello Stato e per le aspettative degli operatori economici e di tanti disoccupati che attendono, soprattutto nel Mezzogiorno, che ciò si realizzi definitivamente. Il mio Gruppo auspica vivamente che il Governo non prosegua su questo tema a far finta di niente, lasciando passare la mozione, sapendo che poi non se ne terrà nessun conto, come accade ormai troppo spesso. La situazione in cui versa il turismo balneare è, infatti, solo uno dei tanti problemi del turismo italiano. Basti pensare allo sviluppo del turismo nel Sud Italia. Il Meridione potrebbe costituire un volano per il turismo italiano, se si volesse davvero sostenerne lo sviluppo tramite i necessari interventi infrastrutturali, un pacchetto di politiche economiche e fiscali orientate agli investimenti, nonché politiche mirate di promozione turistica integrata. Più volte vi abbiamo esortato a farlo, ma siete stati sordi e continuate ad esserlo. Sinceramente - e concludo - quello che abbiamo letto nel nel Documento di economia e finanza relativamente all'istituzione di distretti turistici nel Mezzogiorno, di cui fa menzione anche il testo che ci apprestiamo a votare, non costituisce sicuramente una soluzione per il rilancio del comparto turistico. Ci piacerebbe vedere, invece, che le parole del Senato in questa occasione venissero prese sul serio e che, una volta pubblicamente condivise, vi si desse un seguito. L'Italia dei Valori voterà a favore di questo ordine del giorno per dare un segnale di azione e di vicinanza a quelle imprese che, in un quadro di incertezza e ambiguità, ad oggi restano aggrappate ad una proroga che permetterà loro di lavorare fino al 2015 e dopo non si sa. Queste persone devono avere la certezza che il loro operato in questi anni non è passato inosservato agli occhi del resto del Paese. Infatti, se il turismo è un'industria chiave per l'economia e l'occupazione del nostro Paese e soprattutto - ripeto - per il Mezzogiorno, rappresentando quasi il 10 per cento dell'economia nazionale, dipende anche dalle capacità di queste persone e dal valore di quella ospitalità che questa categoria ha saputo sempre offrire ai suoi clienti.

insieme per dare al Governo, in questo momento di grande difficoltà, la forza di un impegno europeo, che non sarà certamente facile. Nessuno si illuda sarà facile intervenire a livello europeo per estrapolare dall'ambito della direttiva servizi (ovvero direttiva Bolkestein) il settore turistico-balneare, così come noi chiediamo.

che per noi è quasi di principio, ma che difficilmente potrà essere compresa a livello europeo. Per rispondere al collega Pastore, che ha svolto un intervento sulla direttiva Bolkestein chiedendo come sia stato possibile inserire nella direttiva servizi anche questo comparto, che ha la sua peculiarità, la sua specificità

in cui la concorrenza, rispetto all'aumento del PIL in questo settore, è notevole e va considerata come si deve, non fosse altro che per il fatto che ci sono 30.000 piccole e medie imprese che in questo settore hanno investito, che sono a salvaguardia di diversi diritti e

che non sono solo quelli dei gestori di queste aziende balneari, ma anche quelli degli utenti della balneazione, che in Italia sono tanti (tutta la nostra popolazione, dai bambini agli anziani), che devono ricevere un servizio di qualità all'altezza delle sfide dell'attuale turismo globale, che noi dobbiamo assolutamente considerare.

che possano essere recepite; ma soprattutto, va tenuto in considerazione il disposto dell'ordine del giorno G1, che non riguarda soltanto l'articolo 41 della direttiva, ma la possibilità di introdurre una norma in deroga

Sottosegretario, una piccola nota, un tantino meno dolce rispetto a quanto detto prima, ma doverosa.

possibile illegalità o quanto meno di fuori dalla legalità. Credo che essere giusti e rispondere alle legittime aspettative di un settore che merita, perché offre un grande servizio pubblico di qualità e influisce beneficamente sul nostro prodotto interno lordo, per noi sia un dovere,

vi siano sbavature di illegalità, che purtroppo a noi spesso vengono denunciate, in varie parti d'Italia, e non soltanto in alcune Regioni. Infatti, tutto il mondo è Paese, l'Italia è lunga e le deviazioni dalla norma vi sono

condotto con i colleghi di maggioranza e di opposizione, e mi auguro che effettivamente l'Italia possa avere una voce più forte grazie all'unità che il Parlamento oggi ha saputo dimostrare.

con la consapevolezza di ciò che stiamo facendo. Ha ragione la senatrice Sbarbati quando dice che questa unità del Parlamento dà più forza al Governo per aprire una discussione.

Prendo le distanze da alcuni toni, che qui ho ascoltato, di una rivendicazione antieuropea di specificità. Credo che, quando si è discusso questo argomento, probabilmente si è favorita qualche categoria e se ne è sfavorita qualche altra, credo che su questi argomenti dovremo tornare anche per altre categorie, perché il problema si sta affacciando anche per altri. Abbiamo tutelato alcuni grandi interessi in quella sede e sacrificato alcune categorie forse - e sicuramente a torto - ritenute meno significative. Questo è infatti avvenuto. Tra qualche settimana verranno da noi i rappresentanti del commercio ambulante, con lo stesso problema. Non so se il tema della concorrenza nel nostro Paese si debba risolvere partendo dal commercio ambulante o dalle spiagge. C'è quindi un tema più generale ed un tema di certezze. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane

che in queste ore, mentre stiamo parlando, nelle norme sul rilancio dell'economia ci sarebbe anche un intervento sulle spiagge che porterebbe a novant'anni il termine della concessione e quindi renderebbe gran parte di questa discussione superata,

con coerenza di posizioni e con il sostegno di tutto il Parlamento. Ritengo che ciò vada fatto; poi, tra qualche ora, sapremo cosa ha prodotto il Governo su questa materia e cosa si dovrà discutere nei prossimi mesi. La mozione unitaria rappresenta l'auspicio che vi sia unitariamente una revisione della legislazione e delle responsabilità in questo campo. Altrimenti faremo finta di aver realizzato qualcosa e arriveremo al 2015 avendo il problema drammaticamente di fronte a noi.

che sono stati introdotti con questa direttiva. Quindi è molto importante che oggi il Parlamento si esprima in modo unitario per dare forza all'azione del Governo; non sarà facile, ma ci proveremo. Mi auguro che una volta tanto l'Unione dia dimostrazione di non essere sempre quella matrigna che immaginiamo, ma che, entrando nel merito del problema, ci aiuti ad individuare una soluzione che dia garanzia

Signor Presidente, nel motivare il voto del nostro Gruppo, la cui posizione è stata già illustrata dai colleghi Mercatali, Armato e Granaiola,

poi con la legge comunitaria del 2010 ancora all'esame della Camera, con il federalismo demaniale, che poteva essere un'occasione importante per disciplinare meglio tutta la materia delle concessioni demaniali marittime, con gli interventi,

pervenire ad una nuova disciplina nel rispetto certo della trasparenza degli affidamenti delle concessioni, della tutela del patrimonio pubblico, di cui ci siamo fatti carico anche nel passato, della normativa europea e nel contempo della tutela della preziosità

nell'ordine del giorno - la non applicazione della direttiva Bolkestein. Il sentiero è molto stretto e con questo ordine del giorno si chiede al Governo di avviare un negoziato serio, informato, con tutti gli elementi, con l'istruttoria dovuta,

che oggetto della concessione non è un servizio pubblico in senso stretto ma un bene demaniale, un bene immobile - storicamente è così sul quale gli operatori privati gestiscono un servizio privato e fanno un investimento privato che, a conclusione del periodo della concessione, viene acquisito, a legislazione vigente, al patrimonio pubblico. Non sarà possibile uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein all'esito di questo negoziato? Allora si metta mano ad una normativa che tuteli l'interesse pubblico, valorizzando

in modo tale da consentire l'ammortamento degli investimenti in un periodo congruo, magari legando il periodo anche alla quantità e alla qualità degli investimenti medesimi, e ancora tutelando l'avviamento commerciale oppure si rivaluta la possibilità di reintrodurre il diritto di prelazione o di insistenza che è stato criticato, censurato dall'Unione europea, che pure era vigente da molto tempo nel nostro ordinamento. Noi abbiamo presentato non solo questa mozione, ma anche un disegno di legge organico, sul quale hanno lavorato la collega

Non serve un'altra norma transitoria; non si può risolvere questa vicenda con un'altra norma transitoria. il testo dell'ordine del giorno non è preciso. Serve una disciplina stabile e duratura nel tempo, che corrisponda alle esigenze che abbiamo sottolineato e dentro la quale ci può essere lo spazio per una disciplina transitoria, ma all'interno di un quadro di certezze

che indubbiamente dà lavoro, ricchezza, occupazione, benessere e rimane un elemento fondamentale del nostro sistema turistico nazionale, anche rispetto alle sfide di altri Paesi e rispetto all'offerta turistica in generale.

investimenti e l'accesso al credito. In precedenza, come sapete, per quattro anni o, peggio ancora, per un anno, nessun istituto di credito era disponibile a far credito ai titolari delle concessioni. La normativa, nel corso della sua evoluzione, ha definito quindi un quadro oggettivo di certezza. Anche per quanto riguarda il rapporto di locazione, di affitto o di comodato (cioè la cessione a terzi delle aziende),

di cedere ad altri l'utilizzazione della concessione stessa a vario titolo. Si era pertanto arrivati ad un clima di tale certezza del quadro normativo e del rapporto contrattuale che, indubbiamente, ha dato una spinta in avanti al sistema turistico nazionale,

non possiamo dire di non aver lavorato seriamente in questi anni. Abbiamo lavorato più che seriamente perché abbiamo fornito un quadro normativo di una certezza assoluta per quanto riguarda la disponibilità e la utilizzabilità di queste strutture, ottenuto dei grandi cambiamenti in termini di qualità, cambiamenti tali che ci hanno resi fortemente competitivi sul piano internazionale. Poi è arrivata la direttiva servizi che ha cancellato il diritto d'insistenza

Ora, non credo che questa sia una posizione che possiamo accettare con superficialità,

Anche l'indotto viene meno, perché senza l'investimento diretto anche l'indotto non riesce a trovare uno sbocco per i propri servizi e per le proprie merci.

tutto questo debba essere sostenuto, così come purtroppo è stato sostenuto da parte di alcuni soggetti, ma dobbiamo reagire, anche perché abbiamo visto che nei confronti di interessi vitali - in questo caso, economici - del nostro Paese non possiamo chinare la testa e fare finta che nulla sia successo, in relazione a un comparto così importante quale quello dell'offerta turistico-balneare. Giustamente,

un confronto serrato, forte e autorevole, in grado di far capire che per l'Italia questo costituirebbe un danno enorme in termini economici, di occupazione, di sviluppo, ricchezza e competitività.

queste aziende, rischiamo di assistere anche a uno sfratto collettivo di migliaia di famiglie che dovranno essere necessariamente estromesse dall'utilizzazione delle strutture turistico-balneari.

sull'altare di una direttiva che non tiene conto - come è stato già sottolineato - delle particolarità e peculiarità del sistema turistico balneare italiano? Credo che tutto questo vada ben spiegato e fatto capire alle istituzioni europee in quanto - ripeto - non possiamo consentire che il nostro Paese abbia danni così profondi.

per chiudere e risolvere un contratto. Dico tutto questo per citare un altro esempio, ma che comunque rientra nel quadro complessivo delle concessioni demaniali che non può essere assolutamente accettato dal Parlamento.

lo sforzo del Senato, e ringrazio il mio Capogruppo per aver preso l'iniziativa affinché ci sia una nuova normativa che dia certezza a tutti gli operatori di un settore così importante per l'economia del nostro Paese, che è un fatto certamente positivo. Mi auguro che, con una intelligente contrattazione in sede europea, fino a questo momento mancata da parte del Governo, si consideri la specificità del settore.

una adeguata rappresentanza dei diritti dei cittadini di poter usufruire di quel grande bene comune che è il mare e di poterlo fare liberamente, perché in alcuni tratti delle nostre coste ciò non è possibile

di una certa rilevanza. Diritto dello Stato, dicevo, ma anche dei Comuni, se ci fosse sul serio il federalismo demaniale. Mi compiaccio di questo largo consenso, a cui di fatto mi aggiungo, se non fosse per un piccolo passaggio, che ho il vezzo di sottolineare, che non condivido. quella parte dell'ordine del giorno in cui si impegna il Governo «a promuovere l'introduzione di una norma transitoria di lungo periodo». Questo no, colleghi!

Ci sono molti modi per riconoscere il valore residuo degli investimenti, l'avviamento dell'azienda, i mancati guadagni futuri, l'occupazione. Molti modi ci sono, e stati individuati nell'ordinamento: l'unico modo non è quello di rendere la transitorietà eterna.